L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B

In Veneto in questo momento ci sono città allagate, fiumi esondati, strade franate e chiuse al traffico, scuole chiuse, ospedali che stanno per essere evacuati, migliaia di famiglie che hanno subito ingenti danni alle proprie abitazioni e migliaia di ettari di campagne allagati, con notevoli danni all'agricoltura. Le aree comprese tra San Bonifacio, Soave e Monteforte d'Alpone nel veronese, Vicenza e Caldogno nel vicentino e Ponte San Nicolò a Padova sono le più colpite. Come Gruppo Lega Nord Padania chiediamo la massima mobilitazione di tutte le forze possibili per mettere in sicurezza i centri abitati ed occuparsi dei circa 2.500 sfollati che hanno perso tutto, anche la casa. Chiediamo al Governo, che già è prontamente intervenuto, il massimo impegno, da oggi e per i prossimi giorni, a garantire tutto quanto necessario per affrontare al meglio questa drammatica emergenza. al meglio questa drammatica emergenza. Ci sembra giusto, infine, ringraziare chi in questo momento sta lavorando a sostegno delle nostre comunità. Mi riferisco, in particolare, all'Esercito, alle forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, agli enti locali, alle polizie municipali, alla Protezione civile

normalmente si concede alla fine della seduta, per decisione della Conferenza dei Capigruppo, che prevede un'eccezione solo quando la parola è richiesta da un Presidente di Gruppo. Stanti però l'attuale situazione e l'importanza del tema sollevato, credo che brevi interventi, uno per Gruppo, debbano essere in questa fase consentiti.

l'organizzazione ed il coordinamento delle forze istituzionali e dei volontari: era tutto ben preparato. Ma ho visto anche la disperazione della popolazione e dei sindaci, i quali si rivolgono a noi parlamentari tutti, ritenendo che il cordone della borsa - così mi è stato detto - lo teniamo noi: in realtà, è in mano al Governo. Il Governo si era reso presente con il Sottosegretario, ha tenuto riunioni in prefettura a Vicenza e a Verona ha promesso di far dichiarare, entro il più breve tempo possibile, lo stato di emergenza. Ebbene, venerdì si riunirà il Consiglio dei ministri: preghiamo il Governo di ricordarsi questo impegno. In secondo luogo, se il Governo venisse in questa sede a raccontare i fatti a fare un consuntivo, lo preghiamo di fare anche un preventivo, nel senso che prevenire è meglio che curare, anche rispetto all'ambiente, alla vita dei nostri enti locali e dei nostri cittadini.

di ambiente c'è molto da fare: è una priorità che il Governo potrebbe scegliere, e in questa sede troverebbe l'alleanza del Parlamento per individuare le priorità ed i finanziamenti. I sindaci hanno detto che da anni sottolineavano le difficoltà di garantire l'assetto idrogeologico della parte Nord di queste Piccole Dolomiti: c'è un solo torrente che riceve l'acqua da tutti i torrenti ed è di tutta evidenza che, se non viene regolarizzato quello, ci troveremo di nuovo in situazioni simili. Speriamo di no, ma abbiamo avuto i casi della Toscana, della Liguria e della Sicilia: francamente, il Paese merita una priorità assoluta. I sindaci chiedono questo ed ai sindaci dobbiamo dare conto, perché rappresentano le nostre popolazioni. Tutti i volontari e tutte le forze che si sono fatte coordinare dalla Protezione civile meritano davvero un plauso, con l'augurio che il loro lavoro finisca presto, perché purtroppo anche stamattina la situazione a Monteforte d'Alpone era ancora grave. *(Applausi

è stata tale che, nonostante il preallerta della Protezione civile, in alcune realtà e situazioni non si è riusciti a tenere gli argini dei torrenti e l'esondazione è avvenuta, colpendo i territori tra le province di Verona, Vicenza e Padova. questi, signora Presidente, che non sono interessati agli effetti di dissesti idrogeologici: i nostri sono buoni territori e quelle, in particolare, sono zone tutte vocate e dedicate

per aiutare i nostri agricoltori a non patire ulteriori drammi da questo evento. Il prefetto della nostra città, Perla Stancari, ha coordinato nella giornata di domenica l'unità di crisi che poc'anzi il presidente Bricolo ha ricordato, composta dalle forze dell'ordine e di sicurezza, l'Esercito, i nostri Vigili del fuoco e la Protezione civile, per essere vicini ai sindaci ed alle popolazioni che improvvisamente si sono trovati a dover fare i conti con questa realtà

Nel pomeriggio di domenica il sottosegretario Bertolaso era già in contatto con noi, non solo con il prefetto e con la sede della Protezione civile locale, ma anche con i parlamentari che immediatamente hanno richiesto il suo intervento e, tra questi, la sottoscritta.

La nostra attenzione è altissima. Noi chiediamo che il dopo emergenza venga affrontato dal ministro Matteoli

Ritengo che, oltre ai ringraziamenti per il lavoro svolto da chi, anche in termini volontaristici, ha provveduto ad aiutare le nostre popolazioni, ci siano da parte nostra la disponibilità, l'attenzione e l'impegno a sostenere il Governo nell'affrontare il dopo emergenza nel migliore dei modi. Signora Presidente, anche noi ci associamo alle parole dei colleghi di maggioranza e di opposizione che sono intervenuti per esprimere alle popolazioni colpite dalle alluvioni in Veneto, ma anche in altre parti del territorio d'Italia, al Nord, al Centro ed al Sud del Paese. Vorrei fare brevissime considerazioni; anzi, una richiesta e una considerazione. La considerazione è la seguente: gli eventi alluvionali di questi giorni, ove ve ne fosse ulteriormente bisogno, certificano lo stato di dissesto permanente del nostro territorio, dalle Alpi si tratta cioè di tutto il territorio nazionale. Un anno fa in quest'Aula noi abbiamo pianto i morti di Giampilieri e di Scaletta abbiamo continuato poi con un bollettino interminabile di guerra di strade interrotte, di ferrovie dissestate, di treni deragliati e così via. Questa è una vera e propria emergenza nazionale, che arreca un danno economico

purtroppo, si stanno verificando eventi che hanno una loro drammaticità, ancorché fortunatamente un bilancio in termini di vittime limitato. La richiesta che le rivolgo, signora Presidente, è che il Governo venga a riferire in Aula, ma non solo sulla vicenda che possa riguardare il Veneto, ma sull'emergenza e su tutto il bollettino di guerra - chiamiamolo così, impropriamente -che riguarda il nostro territorio nazionale, dal Nord al Sud, per capire che cosa si vuole fare. Altrimenti, stiamo qui ogni mese, ogni anno, ogni autunno a compiacerci del pronto intervento di Bertolaso, della Protezione civile e dei Vigili del fuoco - che non è in discussione e a cui va anche il nostro plauso - della necessità di intervenire tempestivamente con l'Esercito, il Genio militare e così via, della necessità di prevenire con interventi di messa in sicurezza del territorio. Dopodiché, ci troviamo con una legislazione assolutamente inadeguata ,che attribuisce competenze a Comuni, Province, Regioni, allo Stato e, nello Stato, alla Protezione civile, al Ministero dell'ambiente, al Ministero delle infrastrutture e pure al Ministero dell'interno, e non capiamo quali risorse sono a disposizione, come si interviene in maniera strutturale ed organica. Quello che manca fra i tanti piani annunciati da questo Governo - ogni Consiglio dei ministri si deve fare un piano: uno per il Mezzogiorno, uno per la giustizia, uno per la mafia - è un piano di prevenzione, di tutela e di salvaguardia per l'ambiente, che è la vera emergenza che sta mettendo in ginocchio l'economia nazionale. Quindi, chiediamo un'informativa, a 360 gradi, del Governo su tutta la questione che riguarda emergenze, protezione civile e dissesto idrogeologico nel nostro Paese.

abbiamo visto che ormai tutte le Regioni stanno soffrendo il dissesto idrogeologico. Ne parlo con cognizione di causa perché vengo da quel mondo, un mondo dove si studia

sono inermi, perché non c'è una politica di risanamento idrogeologico. Il Governo deve allora intervenire per risolvere questo problema. L'Italia dei Valori ha presentato una mozione a tal fine. Il problema sono le esondazioni, gli argini,

e non solo alla Protezione civile, di realizzare un monitoraggio di tutte le zone a rischio, perché lo sviluppo edilizio è andato oltre la legalità.

Presidente, l'ennesimo evento eccezionale si è abbattuto su un territorio fragile e vulnerabile come il nostro.

onestamente al presidente Bricolo che sarebbe opportuno evitare il regionalismo delle catastrofi, il federalismo delle emergenze.

Peraltro, la prossima Conferenza dei Capigruppo potrà anche prendere in considerazione l'inserimento di questo tema. Abbiamo così esaurito gli interventi sul punto sollevato dal presidente Bricolo.

di studi e di attività che rischiano di chiudere con una norma siffatta. Per cercare di tutelare il lavoro di alcuni avvocati, si mettono di fatto in mezzo alla strada persone che attualmente lavorano, cui è concesso di lavorare per esempio grazie al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: persone e studi che non hanno ordini o albi che li tutelino in questa società delle corporazioni, ma che hanno semplicemente - ripeto,

elettronico, dell'emendamento in esame, e poi parleremo anche delle lettere che arrivano, sperando che qualcuno abbia anche l'intenzione di rispondere.

l'opposizione dell'opposizione, ma quando c'è da fare le leggi per difendere le corporazioni l'accordo con il centrodestra è davvero meraviglioso. Quando si tratta di creare nuovi strapuntini, nuove seggioline, l'accordo con l'Italia dei Valori c'è sempre. Quando si tratta di difendere le corporazioni, l'accordo c'è sempre. Senatori dell'Italia dei Valori, al di là delle indicazioni che vi vengono dal Capogruppo in Commissione giustizia, leggete gli emendamenti che andate a votare, leggete quello che state facendo, perché credo sia utile. Ringrazio invece i senatori

Una consulenza stragiudiziale finalizzata alla stipula di accordi transattivi - il che significa finalizzata ad atti che hanno un valore giuridico e che rientrano nell'ambito di normative è ancora più delicata dell'attività giudiziale, perché si tratta di definire stragiudizialmente rapporti che hanno una ricaduta nel campo del diritto, senza il controllo di un giudice.

Ovviamente, il voto sugli emendamenti di questo disegno di legge non ha un contenuto politico ed ideologico. la libertà di poterci esprimere liberamente, senza farci condizionare da giudizi politici. Stiamo discutendo di un tentativo di riformare la professione forense dopo speriamo di riuscirci. Non sarà un ottimo lavoro, ma ci sforziamo in questa direzione. Quindi non accogliamo lezioni abbiamo libertà e capacità di determinarci liberamente. Voi siete intruppati in una gabbia ideologica.

a chiunque non eserciti la professione in modo continuativo a tempo indeterminato per l'intera vita; cioè stiamo tagliando fuori chiunque si occupi di diritto in modo marginale. Mi chiedo, e chiedo a voi, se questa scelta, che viene compiuta con grande severità, non dovrebbe accompagnarsi quantomeno ad una delimitazione dell'attività di Se questa è la logica della legge, definiamo almeno qual è la consulenza sulla quale vogliamo applicare questa restrizione così drastica. Ieri abbiamo sentito il collega Li Gotti spiegarci che l'atto di querela, cioè l'atto con cui si attiva un procedimento penale in materia di diffamazione

Qui noi legittimiamo ad occuparsi di diritto i non iscritti all'albo, che siano dipendenti di un datore di lavoro, purché lo facciano solo nei confronti di quest'ultimo.

per esempio - al lavoro a progetto, al lavoro cooperativo, al conferimento di lavoro in società, al lavoro in partecipazione, al contratto d'opera (articolo 2222 del codice civile).

Ci si chiede allora «perché» - scrive uno studio - «una attività che si svolge al di fuori delle aule di tribunale debba essere riservata esclusivamente agli avvocati i quali, per loro origine e tradizione, svolgono la loro funzione esclusiva» - giustamente - «all'interno dei tribunali. L'attività stragiudiziale è sviluppata in Italia in maniera onesta e altamente professionale da tantissimi operatori che svolgono da anni il loro lavoro. Se questo articolo sarà approvato, tutti questi dovranno trovarsi un altro mestiere per mantenere le proprie famiglie». Andiamo avanti. «Quello che ci aspettiamo è di poter continuare a vivere e a esercitare la nostra professione onestamente e senza censure in uno Stato dove sia possibile lavorare in un libero mercato, così come accade nel resto dei Paesi europei. Non è neanche lontanamente pensabile, infatti, che in un Paese civile l'assistenza stragiudiziale al di fuori dei tribunali sia riservata esclusivamente agli avvocati. L'articolo 2, comma 6, è contrario ad ogni diritto di civiltà e va contro le raccomandazioni della Comunità europea che vuole favorire, invece, con ogni mezzo, la conciliazione e la composizione bonaria delle controversie. Il nostro accorato appello è teso alla salvaguardia di migliaia di posti di lavoro di professionisti onesti che contribuiscono con la loro attività alla tutela dei diritti dei cittadini italiani, offrendo un aiuto serio e indispensabile. È giusto che anche gli avvocati, come tutte le altre categorie di professionisti, si misurino con un libero mercato, dove la concorrenza per forza di cose sviluppa un servizio sempre più efficiente a tutto vantaggio del cittadino». Il rischio che si corre è che, se l'assistenza stragiudiziale viene fornita e non vi si va poi in tribunale, ciò davvero fa mancare il lavoro anche agli avvocati.

l'attività del serio avvocato è molto più stragiudiziale che non giudiziale e le sue responsabilità sono più forti nel favorire una transazione o una scrittura transattiva, che può dare luogo a nuove incidenze forti nella sfera giuridica dei contraenti) sia un orecchiante, un mestierante,

come tale dev'essere un professionista serio e non l'avvocataccio all'angolo della strada o sotto il lampione, come certo iperliberismo mercatista vorrebbe sostenere in chiave di dottrina professionale. *(Proteste della senatrice Poretti).* Mi dispiace, la filosofia è questa. Quando dite che in Commissione non abbiamo voluto confrontarci, dite cosa falsa: falsa: abbiamo semplicemente e onestamente un'impostazione diversa e democraticamente cerchiamo di farne valere gli argomenti. Tutto qui.

che oggi sono state evocate - lo dico con tono sommesso - un po' a sproposito. Basta leggere il testo che recita: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto

ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata...». In sostanza, si possono instaurare dei rapporti che consentono ad aree vaste del mondo professionale (fatti salvi naturalmente coloro che svolgono attività espressamente regolamentate) di porre in essere tutte quelle iniziative che non siano l'attività legale. Abbiamo limitato quest'ultima agli avvocati, nel solco di un'esigenza fortemente avvertita, ma ci siamo resi conto che per far questo dovevamo determinare un professionista di alto livello. Abbiamo così imposto l'aggiornamento costante e richiesto per la specializzazione corsi continui. Peraltro, abbiamo affidato responsabilità certamente non secondarie - e questo è emerso nel corso del dibattito - a soggetti che avevano la capacità di assolvere a quegli impegni. Vi è poi una serie di altre attività che possono essere realizzate nel quadro di rapporti, anche contenziosi, tesi alla conciliazione, alla sintesi e così via; queste possono essere svolte da soggetti

si ricevono continuamente sollecitazioni, quasi che l'avere individuato requisiti per svolgere determinate e delicate funzioni (quale la consulenza stragiudiziale) sia qualcosa di ottuso rispetto alla modernità dei tempi.

dal comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 711, a prima firma del senatore Casson (pagina 86 del fascicolo),

fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto». Questo è il principio che ha trovato un'esplicitazione più ampia nell'emendamento in esame; noi non ci siamo allontanati

ad un'associazione imprenditoriale di dare consulenza in materia di diritto del lavoro, di diritto industriale o di qualsiasi altra branca del diritto, a soggetti che non siano iscritti all'associazione medesima.

quotidianamente e in modo assolutamente pacifico. Se non è questo che volete, fermiamoci un attimo per pensarci, perché questo è quanto stiamo votando al momento.

un'altra. Come lei sa, il nostro Gruppo ha presentato alcune interrogazioni rivolte al ministro Maroni, al Presidente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri, e ieri in Conferenza dei Capigruppo abbiamo chiesto che il ministro Maroni venga a riferire sulla nota vicenda maturata nei giorni tra il 27 e il 28 maggio.

perché, immaginando che da parte del mio Gruppo potesse intervenire la richiesta (che di fatto era già intervenuta con la presentazione delle interrogazioni) di una sua presenza in quest'Aula, mi faceva presente che avrebbe potuto essere in Senato nella giornata di giovedì, poiché prima era impegnato in una missione in Israele. Ieri, in Conferenza dei Capigruppo, ho fatto riferimento a questa disponibilità del ministro Maroni, frutto di una cortesia - ripeto - personale, ma soprattutto politica e istituzionale

- e mi rivolgo a tutti i colleghi che hanno partecipato alla Conferenza dei Capigruppo - in maniera interlocutoria, poiché da parte delle opposizioni si insisteva perché la disponibilità mostrata dal ministro Maroni di venire in

Chiedo pertanto che il Governo venga attivato con il massimo della pressione possibile, perché il Parlamento della Repubblica non può stare in *stand-by* di fronte alla «melina» giocata su un appuntamento essenziale per la vita politica del Paese, e anche per la sopravvivenza del Governo.

Presidente, il ministro Tremonti ci ha detto che intende inserire nella Costituzione repubblicana il principio per cui tutto ciò che non è vietato è consentito. Se noi volessimo trasferire questo principio nella legge che stiamo approvando, dovremmo scrivere al posto di questo emendamento: «fuori dei casi in cui vi sia un motivo grave di limitazione dell'attività di consulenza, l'attività medesima è libera». il vostro emendamento dice: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge ...», al di fuori di questo caso, la consulenza è sempre vietata. Guardate che per consulenza si intende l'attività

un ordine, un albo, un inquadramento preventivo dell'attività intellettuale dell'uomo in questo campo importantissimo, cioè il campo del diritto, che permea di sé tutta

Avete in mente una società nella quale, sostanzialmente, la cultura viene irreggimentata, viene irrigidita in schemi preconfezionati. È quello che nell'ordinamento corporativo si chiamava «l'inquadramento costitutivo» che è esattamente il contrario di quello che la Costituzione repubblicana ha invece sancito come principio generale di libertà delle attività

gli avvocati stanno mettendosi contro l'intera società civile: «Non so perché gli avvocati e i loro *supporter* in Parlamento abbiano scelto di mettersi tutti contro

sulle proposte 22.201 (testo 2), 28.0.200 (testo 2), 28.0.200 (testo 2)/l, 28.0.200 (testo 39.700, 39.700/1, 41.700, 39.901/1, 39.901/2, 39.901/3,

e 28.700 (testo corretto) in grado di risolvere i profili critici espressi dalla Commissione bilancio rispettivamente sugli articoli 22 e 28. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulle proposte 24.202 (testo 2) e su tutti i subemendamenti riferiti alla proposta 39.1000, nonché parere non ostativo sulle proposte 33.700, 39.901, 16.226, 16.227 e 17.251. Il parere è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni; - che alla proposta 38.200 (testo 2) dopo le parole: "possono stipulare convenzioni" siano aggiunte le altre: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; che alla proposta 38.750, dopo le parole: "apposita convenzione" siano aggiunte le altre: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; - che all'emendamento 39.1000, sul quale il parere è di semplice contrarietà, prima delle parole: "decorso il primo anno" siano aggiunte le altre: "Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato". Resta sospeso il parere sulle proposte 46. 900, 47.1000/2, 64.700 e 66.0.700».

il senatore che ha sottoscritto l'emendamento può ripresentare automaticamente e liberamente l'emendamento riformulato, è un lavoro che non finirà mai. Ovviamente, lo

65 (quello che per l'appunto si occupa della fase transitoria) e non venisse mantenuta in questa parte dell'articolato.

sono dispensati dalla frequenza dei percorsi formativi di cui ai commi 2 e 3 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al comma 3». gli avvocati che all'entrata in vigore della stessa risultano iscritti all'albo da almeno venticinque anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di 2 discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa e significativa esperienza». Cosa significa questa norma? Che soltanto i giovani devono necessariamente specializzarsi. Da ciò discende quindi un particolare onere e

grazia e giustizia ma dal Consiglio nazionale forense. Quindi, il Consiglio nazionale forense diventa arbitro della vita dei giovani avvocati e su di essi cade il peso delle specializzazioni, potendosi gli altri autocertificare

Presidente, proprio questa norma dimostra che non bisogna mai eccedere nel regolamentare materie così delicate e complesse come l'esercizio della professione forense. L'idea che l'avvocatura debba essere una professione che implica e presuppone una alta specializzazione è idea che condividiamo tutti e su cui siamo tutti d'accordo. Che vi sia la necessità di fare in modo che l'accesso alla professione forense sia frutto di una scelta maturata dal giovane collega che si laurea e che vuole fare questo percorso perché convinto, e non perché trovi, nell'esercizio dell'avvocatura, una soluzione di ripiego,

Ma cosa c'entra, con tutto questo, sottrarre dall'obbligo dell'aggiornamento e della specializzazione gli avvocati che hanno dieci o vent'anni di anzianità i quali, addirittura, possono autoproclamarsi, in un'intesa presa con il Consiglio nazionale forense, specialisti di una materia solo perché ciò è legato al decorso del tempo in cui esercitano l'attività professionale?

dietro e farci dire che stiamo approvando una legge - e lo dico da avvocato - a nostra misura, in quanto, a seconda dell'attività professionale esercitata, siamo dispensati noi, e non i giovani colleghi, dall'esercizio della specializzazione. Presidente, non si possono condividere queste argomentazioni: trovo veramente impensabile che un soggetto che abbia per vent'anni esercitato la professione di avvocato che abbia fatto l'amministrativista, il penalista, il tributarista e, quindi, abbia conseguito credito, notorietà ed esperienze,

Mentre per gli avvocati che da dieci anni svolgono la professione è necessario sottoporsi all'esame del CNF, cioè alla verifica della sussistenza di quei requisiti che consentano di attribuirsi il titolo di specialista, dopo vent'anni di professione, ormai, o si è tributaristi, amministrativisti, penalisti e quant'altro, oppure non lo si diventerà più; oppure, se lo si vuole diventare, non avendo una specializzazione particolare, un'attitudine, un impegno e un'esperienza particolari nel settore, si seguiranno le indicazioni che la legge ha stabilito. Quindi, io trovo questa opposizione da respingere e mi auguro vivamente che il collega D'Alia, che stimo moltissimo e che è persona di grande qualità, come avvocato e come politico, voglia riconsiderare la sua opinione.

un avvocato che per alcuni lustri abbia esercitato la sua attività in un ramo del diritto debba

deve essere sottoposto a questa sorta di forche caudine; ma se ha già acquisito sul campo la sua specializzazione, non ha bisogno del titolo.

francamente vorrei contestare il modo e gli argomenti con i quali il senatore Valentino difende il comma 10. Stiamo parlando dell'esercizio di una professione liberale, come molte altre nel nostro Paese Se quello che sostiene il senatore Valentino fosse vero, un medico generico con vent'anni di esperienza, in qualunque momento della sua vita, avendo maturato vent'anni, potrebbe qualificarsi come specialista nell'una o nell'altra

facendo di volta in volta il penalista piuttosto che il civilista o l'amministrativista (proprio per limitarci agli ambiti più conosciuti, seppure più vasti, e che potrebbero contenere all'interno moltissime specializzazioni: ci può essere chi si occupa di penale nell'economia piuttosto che di criminalità organizzata; ma è inutile che ci dilunghiamo), dopo vent'anni di esercizio, se si è qualificato in un settore, non ha bisogno di dichiararsi specialista. Ma l'avvocato del piccolo centro, come tanti ne conosciamo, che tutta la vita ha fatto il civile, il penale, l'amministrativo, il lavoro, l'esecuzione civile, che si è insomma industriato, come può dopo vent'anni autoqualificarsi come specialista? Francamente non capisco. Pongo anche un'altra

della - lo dico tra otto virgolette - "corporazione", non capisco perché dobbiamo sostenere il comma 10, che è soltanto la norma di chiusura di un intero sistema che pone l'obbligo di continuare a studiare, di formarsi e di specializzarsi soltanto ai giovani professionisti, creando quindi un onere incredibile per la loro affermazione professionale, e lascia invece i vecchi avvocati vecchi in quanto con vent'anni di esercizio, al di là dell'età anagrafica - in una condizione di privilegio che non è in alcun modo giustificabile.

sempre e comunque. Ma siccome questa è una norma transitoria ed è una norma che cristallizza alla data di entrata in vigore della legge chi può fregiarsi di questo titolo e chi no, è solo un privilegio per alcuni, odioso.

di questa norma, a mio avviso, non si deve fare una bandiera particolarmente solenne. Stiamo dimenticando, onorevoli colleghi, che questa è una norma transitoria. questa è una norma transitoria. Non è che a regime stiamo prevedendo un privilegio per chi è più anziano. È una norma transitoria, che reca l'espressione «alla data di entrata in vigore della presente legge» e poi tutto quel che segue: dunque è una norma transitoria.

una norma transitoria concede la facoltà non di essere abilitato in esclusiva ad esercitare quel ramo di professione, ma esclusivamente a denominarsi specialista esperto in quella particolare materia. Non è che chi non è specialista non può esercitare la professione in quella branca:

vedrete che tutto questo scontrarsi, se non è proprio pregiudiziale, è un voler scontrarsi su un principio che non è un principio con la «P» maiuscola; quindi diventa pretestuoso. A meno che il relatore non voglia svolgere ulteriori approfondimenti,

emendamento. Il problema è quello che ha esposto la presidente Finocchiaro. Il collega relatore e i miei colleghi del Gruppo potrebbero fare tutti lo stesso sforzo. Il problema è il secondo periodo di questo comma, collega relatore, cioè l'automatismo,

Collega relatore, vorrei suggerire a lei, dall'alto del suo ruolo istituzionale, e ai miei colleghi di fare un passo convergente.

dovrebbe convenire sul fatto che questo primo periodo del comma 10 dà fastidio a più della metà della categoria ma, non si capisce perché, dà un privilegio a molti che invece - e sono la stragrande maggioranza, collega Valentino - non potranno mai subire oppure ottenere privilegi da questo automatismo. Il messaggio che passa, collega relatore, è sempre lo stesso: pochi ottengono un privilegio, non si sa bene nascente da cosa. È vero che ci sono colleghi che per tirare avanti si sono dovuti formare nel corso delle loro delle loro decennali esperienze su più materie (questo è un fatto, non è un'opinione) e che il mero decorso del tempo attribuisce loro una grande grande cortesia, un grande favore. Non è un caso che l'emendamento del senatore Caruso alzasse questo tetto a 25 anni, per restringere maggiormente quella parte, proprio perché

Presidente, l'avvocato Lusi è stato convincente. Non vi è alcun dubbio. Ognuno deve fare il suo mestiere. Collega Lusi, tutto sommato una riflessione ulteriore

«Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non avere riportato sanzioni disciplinari».

al Consiglio nazionale forense, perché lo posso fare, divento specialista e posso fare il difensore di ufficio. Se non ho i dieci anni di professione, ed è il fatto più logico che accade

Non è così.

dell'avvocato di dare risposte al cittadino. Non stiamo costruendo soltanto la figura dell'avvocato. L'avvocato non è il fine di questa legge, è il mezzo, lo strumento attraverso il quale si rende un servizio alla cittadinanza. Questo dobbiamo averlo ben presente. E allora, quando si dice che un avvocato che ha un certo numero di anni può diventare specialista, si ritiene abbia acquisito tutte quelle capacità per offrire al cliente, quindi all'utenza, un servizio. Non c'è una discriminazione

una figura di avvocato che renda un servizio al cittadino.

più di un'ora e un quarto fa la presidente Finocchiaro ha posto un problema. Dalle 16 di ieri la Conferenza dei Capigruppo ha chiesto

La presidente Finocchiaro ha fatto presente di aver avuto un colloquio direttamente con il ministro Maroni, che aveva aderito a tale richiesta. Ebbene, siamo arrivati alle ore 12,15 di oggi,

Senatore Serra, siamo in contatto sia con il ministro Vito che con il ministro Maroni, il quale però in questo momento è all'estero. ho sentito perfettamente quando la senatrice Finocchiaro ha detto di essere stata contattata dal ministro Maroni; nello stesso momento, il ministro Vito invece sosteneva che il ministro Maroni avesse dato disponibilità per martedì pomeriggio. Da lì è nato l'equivoco.

sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo chiedo al Presidente della 5a Commissione permanente, perché non lo capisco.

siamo tanti avvocati in quest'Aula... Mi correggo, secondo alcuni ci sono troppi avvocati in quest'Aula. proprio perché siamo così tanti possiamo confrontare le nostre esperienze personali e chiederci per un momento anche sulla base di quello che i colleghi ci dicono e ci scrivono in questi giorni con un flusso di messaggi pressoché unanime sulla questione quanta parte dei corsi di cosiddetto aggiornamento professionale è davvero utile per la nostra attività e quanta parte, invece, è pura perdita di tempo. che se ciascuno degli avvocati qui presenti dentro di sé fa questa valutazione, dovrà onestamente riconoscere che quella piccola parte dei corsi di aggiornamento che veramente serve è quella che tutti gli avvocati seri farebbero senza bisogno di alcun obbligo o prescrizione. Inoltre, non è una norma come questa che garantisce la frequenza dei corsi veramente necessari. Se le cose stanno così, e se è vero che questa norma è stata originariamente inserita in questo progetto di legge in funzione di filtro,

se c'è un vantaggio nell'essere un Paese un po' più arretrato degli altri, è solo quello di potersi confrontare con i Paesi nei quali le cose funzionano meglio e recepire il meglio della loro esperienza.

siete in grado di citarne uno solo, benissimo, ma se non siete in grado di portare esempi di questo genere nel panorama internazionale, in particolare in quello dei Paesi più civili e avanzati, forse il caso di ripensare questa norma che oltretutto - guarda caso - pone questo onere irragionevole interamente a carico dei più giovani? Infatti, passati dieci anni, passato il termine per la specializzazione, tutti

il problema della formazione continua era avvertito. È vero che in nessun altro Paese europeo esiste una previsione del genere, ma è altresì vero che in nessun altro Paese europeo esiste una produzione legislativa come in Italia. In Italia le leggi cambiano quasi ogni giorno

si deve prevedere e disciplinare o lasciare esclusivamente alla buona volontà? Noi riteniamo che, in nome della tutela dei cittadini, una qualsiasi forma di disciplina e di regolamentazione debba esserci. Se poi la formazione rappresenterà una beffa, oppure una finzione, questa è altra cosa. Noi speriamo che non sia così;

gli avvocati parlamentari, contro il dissenso di metà dell'Aula, e gli avvocati dopo 25 anni d'iscrizione all'albo o dopo il compimento del 60° anno di età.

se da qualche scranno venisse meno demagogia forse risulteremmo più credibili. I giovani da sempre devono sacrificarsi di più perché, essendo ignoranti (in quanto giovani), devono studiare di più: studiano alle scuole elementari, studiano alle scuole medie, si affaticano alle scuole superiori e si devastano di fatica nelle università; poi, nel mondo del lavoro devono farsi strada. I giovani devono studiare, devono applicarsi per tentare di supplire a qualcosa che non possiamo fare per legge. Il peso dell'esperienza che accumula ciascun avvocato nel corso degli anni è forte,

dell'informazione che lei adesso ha dato e cioè che il ministro Maroni verrà in Aula soltanto martedì 9 novembre. Debbo rilevare, naturalmente, che questo, oltre che essere una evidente sottovalutazione della gravità di quanto sta accadendo oggi nel nostro Paese da un punto di vista sia giudiziario, che delle cronache che occupano praticamente tutti i quotidiani d'Italia e direi anche d'Europa, è anche l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Infatti, tenere il Parlamento all'oscuro di una posizione del Governo su quel che sta succedendo è molto grave. Approfitto anche per chiederle di suggerire al ministro Maroni, visto che per sua iniziativa verrà martedì e non oggi, come avrebbe dovuto, di prepararsi anche a rispondere ad altro, oltre che alle questioni che hanno riguardato la questura di Milano, come lei adesso ha annunciato, quindi a tutto quello che sta accadendo ora e che accadrà da ora a martedì. *(PD)*. Di questo dovrà venire a parlare martedì prossimo, non soltanto della questura di Milano. Presidente, penso che obiettivamente il Governo poteva venire a riferire in Aula anche giovedì mattina prima di concludere i nostri lavori. Non capisco la ragione per la quale si debba prendere tempo. Prendiamo atto comunque che questa è la data fissata, anche

di chiedere a sua volta, per il tramite della polizia, al Ministro dell'interno - perché credo che questo sia stato il giro per riuscire a partorire quella data - di disporre anche una informativa sui provvedimenti di espulsione che eventualmente, al compimento della maggiore età, siano stati adottati nei confronti di extracomunitari che non si trovino in posizione regolare o che siano sotto procedimento penale. Non vorrei che - lo dico a tutela dei colleghi della Lega - in questa circostanza specifica o in altre vi possano essere disparità di trattamento, che sarebbero oggettivamente irriguardose.

sta più a cuore il «caso Ruby», chiamiamolo così, anche se è stata già ampiamente chiarita sia dalla questura che dalla prefettura di Milano

o martedì prossimo. Cambia tanto invece nei confronti degli alluvionati vedere un Parlamento unito che chiede aiuti al territorio, nel momento in cui ci sono 2.500 sfollati, migliaia e migliaia di ettari di campagne allagate, con danni incalcolabili per l'agricoltura, nel momento in cui ci sono strade strade franate, scuole chiuse ed ospedali trasferiti. Questo forse era più importante per i cittadini e andava nell'interesse del Paese. Prendiamo atto dei vostri interventi e andiamo avanti con i lavori dell'Assemblea.

per i toni che sono stati usati. Lei è sempre cortese, direi proverbialmente cortese. Ma in questo caso ho sentito un'aura di minaccia incombere sul ministro Maroni, reo di non essere arrivato tempestivamente,

settori ufficiali della vita istituzionale milanese, perché sia a conoscenza di vicende che gli altri ignorano, che non appaiono sui giornali e che debbono creare questo clima di tensione. Mi auguro vivamente che nell'esuberanza oratoria abbia detto qualcosa che non pensava.

ognuno dei canali privilegiati di cui dispongo io. ci sono dei momenti in cui sicuramente il rispetto delle istituzioni impone al Parlamento una particolare attenzione

A Castelletto Ticino, in Provincia di Novara, è in corso una situazione drammatica per 120 cassa integrati dipendenti dell'ex Imit. La corte d'appello di Torino ha respinto il concordato antifallimentare, che stabiliva tempi e modi per quanto riguarda il TFR dei lavoratori, sia dei cassaintegrati che degli oltre 120 dipendenti riassunti da Imit.

in merito ai danni provocati in alcune zone del Veneto a causa del maltempo che si è lì abbattuto negli ultimi giorni. A tal riguardo è doveroso, da parte mia, segnalare anche alcune zone del mantovano che hanno subito notevoli danni a causa dell'esondazione del fiume Chiese. In modo particolare, il Comune di Asola, che attualmente conta 300 sfollati, soccorsi adeguatamente dalla Protezione civile,

Per il forte disagio subito dalla popolazione di Asola ho già presentato un'interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, interrogazione alla quale sollecito una risposta in breve tempo. Il Gruppo della Lega Nord chiede al Governo di riferire quanto prima in Aula e di assumersi l'impegno a supportare tutte le popolazioni colpite dalle alluvioni, anche quelle colpite nel mantovano. In modo particolare, vorrei che nel prossimo Consiglio dei ministri Un particolare riconoscimento e ringraziamento va, oltre che alla Protezione civile, alle forze dell'ordine, al volontariato, agli enti locali e ai Vigili del fuoco che nel mantovano hanno saputo far fronte all'organizzazione dei primi soccorsi. Ora, è necessario dare sostegno e risposte concrete ai sindaci e ai cittadini colpiti.

sospeso le rate dei mutui da aprile 2009 sino a dicembre 2009 e poi - con un accordo tra ABI e Governo - da gennaio 2010 fino a giugno dello stesso anno. Su quelle rate congelate non dovevano decorrere gli interessi. Ci sono persone che hanno perso la casa e che pagano il mutuo sulle macerie.

oltre alle rate che sono state congelate applica interessi che eccedono di oltre dieci volte il tasso soglia fissato dalla legge 8 Faccio un esempio: dal 30 aprile 2009 fino al 31 dicembre 2009 scattavano interessi di 2.710,38 euro. Invece di calcolare gli interessi semplicemente per quei nove mesi, sono stati calcolati per l'intero ammontare del mutuo, che era di 126.000 euro. Si arriva quindi ad interessi TEG, tasso effettivo globale, pari al 279,99 per

continuare a speculare. Ho già presentato numerose interrogazioni: ieri c'è stata una risposta in Commissione finanze, che non è soddisfacente. Oggi, insieme al collega Mascitelli, presenteremo un'ulteriore interrogazione con fatti concreti.

Cosa è successo? Una delle prove riproduceva esattamente un'esercitazione già effettuata dalla scuola «Anselmo Anselmi» di Roma poche settimane prima e molti dei candidati avevano frequentato quella scuola. Il terzo giorno del concorso alcuni candidati sono stati trovati con la traccia

seduta al vice presidente Chiti. Oggi lo rinnovo a lei. I direttori delle testate a rischio di chiusura, a causa della mancata riproposizione del fondo dell'editoria e del taglio delle tariffe agevolate